degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Una riforma particolarmente attesa e rilevante sia per gli ambiti coinvolti, stante la lunga tradizione italiana nella tutela del patrimonio, sia per l'attenzione mediatica che ha suscitato. Lei stesso Ministro è intervenuto l'11 dicembre 2014 in 7a Commissione cultura e istruzione del Senato per illustrare la riorganizzazione del Ministero, nel suo primo giorno di entrata in vigore. La riforma, ispirata ai principi di *spending review*, affronta per la prima volta questioni annose e strutturali, sulle quali noi concordiamo molto. La *ratio* che ha portato alla riorganizzazione è stata quella di integrare pienamente di semplificare l'amministrazione periferica, di ammodernare la struttura centrale, di rilanciare le politiche di innovazione e formazione, di valorizzare le arti e l'architettura contemporanee con particolare riferimento alle periferie urbane, punto questo molto curato, e di dare maggiore autonomia

(che mi risultano in parte esserci) derivanti dalla mancanza di personale amministrativo non tecnico (perché sulla parte tecnica vi sono state delle assunzioni, di cui sono a conoscenza), nonché del raggiungimento degli obiettivi che tale riforma si era prefissata.

unitarietà del sistema, di trasparenza, efficienza e, soprattutto, di responsabilità, nel senso che si chiarisce bene chi deve fare cosa. Ripeto, però, che non si tratta di una riforma nata dal basso attraverso un confronto pubblico e politico e attraverso un coinvolgimento di tutti i protagonisti in campo. Si tratta di un regolamento e come tale va anche valutato. Vorrei capire esattamente cosa sta accadendo nei 20 musei *top* che sono stati indicati da questo regolamento e le cui nomine sono state fatte da lei e dal direttore generale Soragni. Per esempio, il Museo nazionale romano, che credo sia stato messo a bando, non si sa neanche come si chiami e mette insieme quattro musei: Palazzo Altemps, la Crypta Balbi, le Terme e Palazzo Massimo. Vorrei sapere se i parchi archeologici hanno una normativa di riferimento. Qui a Roma, il Parco dell'Appia antica è anche un parco naturalistico regionale, quindi bisognerà trattare anche, credo, con il Presidente della Regione e capire esattamente quali siano le competenze del futuro parco archeologico. I segretariati regionali fanno coordinamento con le Sovrintendenze? E le Sovrintendenze sono dei corpi isolati? Fanno tutela? I direttori dei musei lavorano con i soprintendenti o sono solo delle monadi, delle isole, dei domini, dei protettorati, cioè quello che il regolamento voleva superare? Noi dobbiamo chiarire tutti questi passaggi perché vedo

Signor Ministro, lo scorso 24 marzo è stato firmato il decreto ministeriale relativo alle modalità di selezione di nuovi funzionari. Dai bandi pubblicati per le assunzioni al MIBACT, risulta che alle biblioteche siano destinati solo 25 funzionari, fatto che decreterebbe la scomparsa collaterale di molte strutture. I fondi supplementari messi a disposizione dal Ministero rischiano di rimanere un provvedimento tampone e privo di efficacia, in assenza di un quadro organico di rilancio del comparto. Com'è noto, il blocco del *turnover* ha causato un sensibile deterioramento dei servizi erogati dalle biblioteche che già al momento sopravvivono con il ricorso al volontariato, tirocini e servizio civile mentre molti giovani professionisti dei beni culturali sono costretti a trovarsi una diversa occupazione spesso dequalificata. La situazione è talmente grave che in segno di protesta i membri del comitato tecnico-scientifico per i beni e gli istituti culturali e il professore Giovanni Solimine del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici hanno rassegnato le dimissioni precisando che in questa situazione, mentre da un lato appare in serio pericolo l'effettivo esercizio da parte dello Stato delle delle funzioni di tutela sui beni librari, lo stesso futuro di molte principali biblioteche del nostro Paese risulta irrimediabilmente compromesso e fortemente pregiudicata la possibilità per esse di continuare a poter erogare un adeguato servizio al pubblico e a favore dell'intera comunità nazionale. Alla luce di quanto esposto, si chiede al Ministro quali iniziative intenda assumere sia per sanare una situazione indiscutibilmente gravissima sia per garantire l'attività del comitato e del Consiglio.

avevano implicito anche l'obiettivo della riduzione dei tempi di risposta e la riduzione dei passaggi amministrativi nelle pratiche ricadenti nell'ambito delle competenze delle Sovrintendenze stesse. Non va sottaciuto che talvolta pratiche complesse per le quali era prevista l'espressione di un parere di diversi settori delle Sovrintendenze, andavano incontro a pareri non sempre uniformi con la conseguente complessità di gestione amministrativa delle pratiche e, per il comune cittadino, di una cattiva concezione della pubblica amministrazione. Si chiede se siano stati effettuati dei monitoraggi sulla effettiva riduzione delle tempistiche oppure se vi sia l'intenzione di farli e se, considerate anche alcune recenti modifiche normative, si possa effettivamente parlare di riduzione dei tempi e di semplificazione delle procedure per quanto di competenza delle Sovrintendenze.

personale per adeguarlo alle previsioni di legge, è stata ridotta la pianta organica di legge per adeguarla alla situazione di fatto. La situazione è destinata ad aggravarsi, se prendiamo in considerazione il numero dei pensionamenti: circa il 60 per cento dei funzionari attualmente in servizio al Ministero dei beni e delle attività

In questo frangente è stato approvato il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che ha sottratto alle Regioni e assegnato allo Stato la competenza in materia di tutela del patrimonio bibliografico,

In tale contesto, nonostante i fondi aggiuntivi previsti attualmente per le biblioteche pubbliche statali, è necessario chiedersi se nell'ambito specifico delle dotazioni organiche di tali fondamentali istituzioni, il Ministro abbia reale contezza dell'attuale situazione, anche attraverso una stima dei pensionamenti dei bibliotecari nei prossimi anni, in modo da valutare l'opportunità di avviare un piano pluriennale di assunzioni che, a differenza dell'attuale concorso per funzionari del MIBACT, il quale prevede su 500 posti soltanto 25 riservati ai bibliotecari, risolva l'attuale situazione drammatica.

dal Ministro interrogato quali saranno le conseguenze e gli effetti del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni, delle attività e del turismo, con particolare riferimento ai cosiddetti nodi ancora da risolvere e alle linee di azione previste e allo scopo implementate, fornendo informazioni volte a conoscere lo stato dall'arte nell'opera di riorganizzazione del Ministero stesso. Signora Presidente, signor Ministro, il nuovo schema di riorganizzazione del MIBACT prevede di adottare un nuovo modello di organizzazione del sistema di tutela del patrimonio culturale italiano, che non prevede più l'esistenza di Sovrintendenze specificamente dedicate all'archeologia nelle diverse Regioni, ma Sovrintendenze uniche con competenze miste distribuite sul territorio su base interprovinciale. Le procedure di tutela si sono sviluppate da decenni separatamente nei diversi settori di competenza tecnica (archeologia, architettura e arti), considerando le peculiarità proprie di ciascuno di essi. dunque le decisioni strategiche in questa materia a dirigenti - anche se coadiuvati da funzionari specialisti - che non abbiano una precisa coscienza della disciplina archeologica, può comportare il rischio di una sottovalutazione delle problematiche di conservazione, con conseguente impatto sui tempi e sui costi degli interventi di archeologia preventiva. La frammentazione delle funzioni di tutela tra più uffici territoriali di dimensioni ridotte rischia di privilegiare un atteggiamento che non consente una visione di carattere generale delle problematiche storiche. Questi nuovi orientamenti organizzativi svalutano il carattere tecnico-specialistico delle Sovrintendenze e ne riducono la portata territoriale alla dimensione provinciale e non più regionale. quindi se il Ministro intenda rivalutare la possibilità di un'opzione interregionale, rispetto alla dimensione provinciale, visto che questi enti sono in fase di ridimensionamento a livello amministrativo generale e se saranno salvaguardati in maniera adeguata, nel nuovo progetto organizzativo posto in essere dal MIBACT, l'interesse alla tutela del patrimonio archeologico e del paesaggio culturale e la continuità dell'azione amministrativa, al fine di evitare che nel lasso di tempo necessario per organizzare la nuova articolazione il territorio italiano, già fragile e sottoposto a numerosi interventi, abbia a risentire in modo irrecuperabile della trasformazione delle articolazioni territoriali del Ministero.

dell'archeologia. In particolare, la riforma Franceschini sugli assetti organizzativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché degli enti vigilati, è arrivata ad appena un anno di distanza da un precedente e controverso intervento di "ristrutturazione" degli uffici e delle competenze, che già aveva causato enormi disagi e, spesso, la paralisi delle attività istituzionali, separando la tutela e la valorizzazione, finora fasi inscindibili di un unico processo. Le Sovrintendenze hanno perso lo sbocco naturale, quello della fruizione delle ricerche sul campo che caratterizzano le attività di salvaguardia. In particolare va stigmatizzata l'abolizione delle Sovrintendenze archeologiche che, come ad esempio quella di Taranto, istituita centodieci anni fa, costituiscono un organo tecnico-scientifico di ricerca dello Stato

e non attraverso modifiche legislative, ma ciò è potuto avvenire per norme specifiche che in due occasioni diverse hanno consentito che l'intervento sulla riforma organizzativa del Ministero avvenisse attraverso norme non di legge. Non penso che le riforme debbano avvenire soltanto attraverso disposizioni legislative: ci sono vari strumenti, dai decreti legislativi ai regolamenti che attuano

che aveva insediato una commissione presieduta dal professor D'Alberti, che ha lavorato per più di un anno e mezzo. In questo caso c'era anche una coincidenza politica, ma anche quando tale coincidenza politica non c'è, penso che non ci sia niente di più sbagliato nel fatto che chi arriva a guidare un Ministero ignori tutto quello che hanno fatto i predecessori e ricominci da capo.

In passato il nostro sistema museale, unico al mondo per qualità e quantità delle collezioni, non è stato oggetto di un investimento vero in termini di modernizzazione e di valorizzazione, in buona parte perché i nostri musei statali - è bene che il Parlamento ne abbia la piena consapevolezza sostanzialmente fino a questo intervento non esistevano. Evidentemente esistevano come collezioni, ma non giuridicamente, nel senso che erano semplici uffici alle dipendenze gerarchiche della Sovrintendenza territorialmente competente. Ciò valeva anche per i grandi musei

più dipendenti dalle Sovrintendenze, ma dalla direzione generale musei e da dei poli regionali museali che hanno il compito esclusivo di investire sulla valorizzazione; le Sovrintendenze, invece, continueranno ad occuparsi di tutela del territorio.

(archeologi, architetti o storici dell'arte) che abbiano anche maturato esperienze di gestione di un museo, che non è la stessa cosa che fare tutela sul territorio attraverso una Sovrintendenza. Già nel primo *step* della riforma,

erano divise in tre settori: archeologia, beni artistici e beni architettonici, spesso con competenze territoriali diverse. Per come si è venuta formando in modo disordinato la mappa geografica sul territorio, nella stessa città potevi avere un bene

Il cittadino farà un'unica domanda e riceverà un'unica risposta e anche i conflitti, che è

(Pompei e Roma). Per il personale - mi è stato chiesto da diversi interroganti

conoscete molto bene perché le ha approvate il Parlamento. Nella legge di stabilità dell'anno scorso è stata introdotta in deroga - c'è un riconoscimento importante di un ruolo dei beni culturali - la possibilità di assumere - il bando è aperto - 500 persone per le professionalità di cui il Ministero era privo da anni per i pensionamenti. Si tratta di architetti, archeologi, storici dell'arte, bibliotecari, archivisti, demoetnoantropologi.

che, dal punto di vista generale, esiste tra i 770 posti vacanti e i 500 posti a concorso. Così si sono determinati i numeri, che

90 archeologi su 136 carenze, 130 architetti su 198 carenze, 95 archivisti su 146 carenze, 40 storici dell'arte su 61 carenze, 30 funzionari della promozione e comunicazione su 50 carenze. Da qui deriva il numero dei bibliotecari,

sul modello di altri istituti, come l'Istituto centrale del restauro, che sarà il luogo in cui raccoglieremo la conoscenza, il *know-how* e le eccellenze, in Italia e nel mondo. L'Italia, infatti, è il Paese che ha più missioni archeologiche

un'attenzione particolare alla questione del personale del Ministero, anche perché abbiamo tantissimi giovani disponibili; anzi, assolutamente intenzionati a inserirsi in questi filoni professionali. Quindi, per noi diventa un dovere offrire loro opportunità.

questo discorso può farlo chi avvia e promuove il regolamento, ma è passato quasi un anno: cosa hanno combinato questi 20 direttori? Hanno fatto una raccolta fondi? Fanno tutela? Vi ricordo che negli Uffizi c'è Botticelli, Michelangelo, Raffaello; c'è il palazzo, ci sono i depositi. Stanno lavorando anche sul fronte della tutela. Tutela significa anche valorizzazione. Diceva Spadolini, tutelare valorizzando e valorizzare tutelando: sono due facce della stessa medaglia. Se lei leggesse la legge Croce del 1922 e le due leggi Bottai del 1939 si accorgerebbe che la valorizzazione - si parlava di valorizzazione anche allora,

Ministro, purtroppo non sono soddisfatta della risposta ricevuta, perché, pur comprendendo che lei sia venuto qui e ci abbia parlato del metodo che ha deciso di adottare, sarei aspettata una risposta più articolata su questo punto, perché comunque le dimissioni di tutti i membri di un comitato così importante hanno provocato uno terremoto accademico. Non si era mai visto, infatti, l'utilizzo di metodi così

con una risposta più articolata, che potesse darci spunti anche sulle direttive di un quadro organico di rilancio del comparto. Invece lei ha fatto spallucce e ha riversato la responsabilità sul Parlamento, auspicando che lo stesso nel corso della prossima legge di stabilità, possa aumentare i posti disponibili. Certo, lei non può, però poteva venire intanto a illustrare - casomai - una qualche linea di indirizzo, una qualche proposta (che non ho sentito). Forse il disinteresse nei confronti del comparto delle biblioteche è dato anche dal tempo relativamente breve che lei ha dedicato alla risposta su questo punto... rispetto invece ai temi più generali posti dagli altri colleghi. Pertanto non sono per nulla soddisfatta. PRESIDENTE. Mi scuso, ma abbiamo tempi molto rigidi. Lo faccio solo per questo, altrimenti sarebbe molto interessante dilungarsi.

Ministro, la carenza di personale cui ha fatto riferimento nel suo intervento ha come parametro il decreto ministeriale del 6 agosto 2015. Tuttavia, ricordo che in quell'occasione la pianta organica era stata già ridotta notevolmente rispetto al 1997 e, già allora,

delle piante organiche, per poi mettere in campo la redistribuzione sulla base dei 500 posti. In conclusione, la ringrazio per la risposta, ma - ovviamente - non sono per niente soddisfatta, perché questo vuol dire aprire, ancora una volta, alla precarizzazione e allo spreco di denaro pubblico.

parzialmente soddisfatto per la seguente ragione. Lei conviene con me che l'archeologia è uno specificità e una tradizione tutta italiana. Giungiamo però a considerazioni finali diverse. Sono parzialmente soddisfatto perché il suo intervento

Signora Presidente, onorevole Ministro, dopo un periodo di crisi il turismo è in forte ripresa in Italia. Certo, bisogna sempre pensare da dove si parte e ricordare,

essendo stati staccati quasi 7 milioni di biglietti (6,6 milioni, per l'esattezza). Si tratta, quindi, di un incremento rispetto all'anno precedente di oltre un milione di biglietti. Il Colosseo è veramente l'epicentro del turismo culturale di Roma, che è la capitale di tutti gli italiani, dal Nord, passando per il Centro,

e di tante altre iniziative; parliamo di fiscalità di vantaggio, fortunatamente, e di mecenatismo moderno. Vorrei sapere anche a che punto siamo con la realizzazione del centro servizi per l'orientamento alla visita e per la gestione 6 milioni di visitatori del Colosseo, che oggi sono costretti a lunghe ed interminabili file, in condizioni di ospitalità, di accoglienza e di orientamento al pubblico veramente indecorose.

Signora Presidente, signor Ministro, il turismo culturale si sviluppa nei luoghi della cultura. I piccoli musei, non per le loro dimensioni fisiche, ma per il modo di intendere il concetto stesso di museo, sono un esempio di veicolo privilegiato del turismo culturale. Sono chiaramente diversi dai grandi musei per la loro specificità, ma anche e soprattutto per il loro rapporto intenso e più stretto con le comunità locali, che li lega indissolubilmente alla storia dei luoghi. Esistono eccellenze nazionali, esempi di grande pregio, come il Museo del Bisso di Sant'Antioco, che sono stati quasi dimenticati o, nella migliore delle ipotesi, non riconosciuti tali dalle istituzioni locali. Mi chiedo come mai spesso questi esempi di arte, di cultura e di tradizione ancora viventi non vengano sufficientemente valorizzati, a partire dal concetto stesso di piccolo museo, inteso come fucina di cultura ed espressione dei territori e delle loro identità, considerate le loro potenzialità, in grado di attrarre turisti da tutto il mondo. Vorrei sapere perché questi speciali e privilegiati veicoli della cultura non vengano sufficientemente riconosciuti con investimenti consistenti, al momento ancora troppo modesti, e politiche di promozione turistica. È possibile

signor Ministro, il decreto legge n. 83 del 2014, contenente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio dei turismo», molto frequentemente è definito e conosciuto come *art bonus* per aver introdotto, in modo sicuramente innovativo in Italia, il concetto di mecenatismo nell'arte. Esso è da ricordare tuttavia per un altro importante aspetto, quello di associare la cultura al turismo. In quest'ottica il turismo culturale, un turismo evoluto (anche dal punto di vista della capacità di spesa), può acquisire una dimensione fondamentale per una nuova fase di sviluppo del nostro Paese. Può sembrare retorica ricordare come l'Italia sia universalmente conosciuta per la grande ricchezza culturale che la caratterizza: siti culturali quali beni monumentali, musei, aree archeologiche, luoghi di spettacolo, luoghi di pregio ambientale, siti UNESCO, centinaia di *festival* musicali, stagioni concertistiche, d'opera, teatrali, iniziative culturali di vario genere, tradizioni che animano i territori. Questa eredità rappresenta non solo il passato e il presente, ma anche il futuro del Paese, una risorsa da tutelare e valorizzare, che ci rende unici nel panorama internazionale. ormai ampiamente noto come non sia sufficiente possedere beni di tal genere; attraverso la loro conservazione ed il loro recupero si deve affermare pienamente il concetto di valorizzazione, anche attraverso iniziative di attrazione turistica. In quest'ottica, di sicuro interesse è anche la direttiva ministeriale sui cammini, che tende ad ampliare l'offerta turistica diffondendo la conoscenza degli itinerari escursionistici pedonali e ciclabili, un tema nuovo per l'Italia, ma molto più diffuso in altri Paesi. A questo proposito, chiedo se sia pensabile che l'applicazione dell'*art bonus* possa avvenire anche per interventi a favore delle iniziative culturali e quali ulteriori iniziative intenda promuovere il Ministero, anche alla luce del fatto che, al di là delle importanti ricadute di tipo economico, la divulgazione della cultura, dell'arte e dell'amore per il bello può contribuire al miglioramento della qualità della vita e prevenire in definitiva anche situazioni di disagio sociale, che portano spesso a conseguenze drammatiche. Presidente, signor Ministro, il nostro patrimonio culturale e turistico rappresenta un'importante opportunità per il nostro Paese. Tuttavia ad oggi in parte in parte queste potenzialità non sono sfruttate. La rivoluzione digitale ha trasformato l'industria del turismo e il *web* si sta affermando sempre più come un luogo di informazione e intermediazione turistica. Nel contesto internazionale, il turismo italiano vive una situazione di decrescente competitività dovuta alla concomitanza di criticità strutturali e fattori congiunturali connessi con la crisi economica. Nell'epoca della globalizzazione e dell'annullamento delle distanze, il tema dell'accessibilità, considerata sia sotto il profilo della mobilità e dei trasporti, ma soprattutto anche per quanto riguarda la rete digitale, divide il Paese in due, ponendoci di fronte un'Italia accessibile ed una inaccessibile. Visto che l'attitudine e i comportamenti dei viaggiatori sono sempre più *social* e *digital*, la promozione digitale rappresenta uno degli *asset* di sviluppo del turismo italiano. Consideriamo che l'85 per cento delle imprese chiuse a livello globale nel 2015 erano aziende prive di un sito Internet. Consideriamo inoltre che il documento dell'AGID «Strategia per la crescita digitale 2014-2020» propone diverse azioni da mettere in campo per risolvere le criticità emerse nel settore turistico, legate al ritardo tecnologico e informatico del Paese, tra cui il potenziamento della Rete, lo sviluppo di strumenti di *marketing* avanzato, la promozione telematica dei *brand*. Si chiede cosa intende fare in proposito il MIBACT per rendere attuative queste indicazioni, che tipo di risorse pensa di investire e con che tempi, visto che ormai ci avviciniamo quasi ad essere «nel mezzo del cammin di nostra vita». Signora Presidente, il piano cultura e turismo approvato recentemente dal CIPE stanzia 1 miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per la realizzazione di innumerevoli interventi di tutela e e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale. Vorrei avere dal Ministro interrogato un approfondimento sui contenuti del citato piano, citato piano, illustrando le principali iniziative per la promozione del turismo culturale in Italia, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di valorizzazione di antichi tracciati e di veri e propri percorsi tematici, volti

il miliardo di viaggiatori, con le classi medie dei Paesi emergenti come Cina, India, Russia e Brasile che premono sull'offerta. L'Italia è comunque nell'Eurozona il primo Paese per numero di pernottamenti

anche le «società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche».

Detto ciò, il nostro Paese in questo momento è al sesto posto, non al quinto, dietro Stati Uniti, Spagna, Francia, Cina e Macao, per quanto riguarda il *business*. Abbiamo più siti UNESCO di tutti gli altri Paesi messi insieme, ma il Louvre da solo stacca più biglietti di tutti i musei italiani messi insieme. Tra il 2015 e il 2016 qualcuno dice che i nostri alberghi hanno registrato

Turchia, Tunisia ed Egitto. Di conseguenza, i nostri connazionali scelgono di rimanere in Italia e per questo motivo qualcuno si riempie la bocca. Si domandi, invece, Premesso questo, signor Ministro, nei mesi scorsi il CIPE ha varato il Piano cultura e turismo, stanziando un miliardo di euro del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per la realizzazione di numerosi interventi su tutto il territorio nazionale, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e per

anche sotto il profilo occupazionale. Camminiamo su giacimenti immensi di reperti, rovine, ritrovamenti archeologici, artistici e architettonici. Ci muoviamo in un paesaggio che è un *mix* singolare, quando non deturpato, di naturale e costruito. Fuor di metafora: l'Italia come "grande bellezza". Tale tipologia di turismo, inoltre, si caratterizza per una maggiore sostenibilità rispetto al cosiddetto "turismo di massa", che incide negativamente sull'uso del paesaggio, del suolo, dell'ambiente. Il turismo dei luoghi e dei beni culturali, inoltre, permette di valorizzare uno degli assetti più importanti di cui l'Italia sia in possesso: la cultura intesa come patrimonio (*cultural heritage*) e di produzione culturale e di contenuti materiali ed immateriali. Per queste ragioni, riteniamo necessario che il Governo avvii delle politiche volte, non solo a consolidare il comparto nella sua interezza, ma che si prodighi nella definizione di politiche volte a sostenere un sempre più intenso ingresso nel mercato di *player* in grado di aumentarne i livelli di competitività e in grado di raggiungere segmenti di domanda nuovi, come il *fashion* e l'enogastronomia. A nome dei Conservatori e Riformisti, chiedo di sapere se il Governo intenda promuovere, e in che tempi, misure fiscali per favorire la promozione del settore turistico-culturale, anche attraverso l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per il turismo culturale e più in generale per la produzione di contenuti culturali.

relativi al turismo nel nostro Paese. Questo perché, alla crescita costante, che è continuata anche negli anni della crisi, del turismo internazionale nel nostro Paese si è aggiunto anche un ritorno del turismo interno.

I Paesi che attraggono turismo internazionale crescono enormemente, cresce la competitività: chi avrebbe detto dieci anni fa che Dubai, in pieno deserto, sarebbe diventata una delle mete più attrattive per il turismo internazionale?

il primo Paese europeo per turismo extraeuropeo. E questi numeri cresceranno fortissimamente. Dobbiamo pertanto mettere a punto delle strategie, ed è quello che stiamo cercando di fare con il Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia che ha avuto già due tappe importanti a Pietrarsa. un meccanismo molto partecipato: abbiamo coinvolto tutte le Regioni, i Comuni, le associazioni di categoria, i privati e il mondo digitale perché esca un piano strategico che alla fine sia condiviso. Poi ognuno farà la propria parte, il pubblico, il privato, lo Stato e la Regione, ma deve essere un progetto condiviso, quindi scritto insieme. Il 27 luglio seduta del comitato permanente per il turismo. Vedremo se sarà quella in cui verrà approvato il Piano strategico per i prossimi cinque anni o se sarà a settembre; dopodiché andrà in Consiglio dei ministri perché questo prevede la legge.

andranno tutti a vedere il Ponte di Rialto, la Fontana di Trevi e gli Uffizi, quei luoghi non ce la faranno. Non ce la fanno già oggi tanto è vero che si parla di *ticket* e di biglietti di accesso perché sono luoghi fragili che possono contenere un certo numero di persone e non un numero infinito. E il paradosso è che in quelle stesse città, o in città a qualche chilometro di distanza, per non parlare del Mezzogiorno e di altre parti d'Italia, ci sono luoghi meravigliosi che in un altro Paese sarebbero da soli in grado d'attrarre turismo internazionale e che non sono valorizzati come meritano. l'Italia come museo diffuso. Quando andiamo a fare promozione all'estero non andiamo a promuovere chi non ne ha bisogno ma le città minori. La stessa idea della capitale generale della cultura che sta avendo un grande

regionali hanno esclusivamente questo compito: valorizzare tutto il sistema dei musei minori statali, perché parliamo di quelli di nostra proprietà, e lavorare per costruire piani di promozione totalmente integrati, almeno con gli altri musei pubblici. Ormai da un anno e mezzo abbiamo istituito un tavolo che lavora con l'ANCI perché davvero, quando un turista arriva in una città, che il museo sia del Comune o dello Stato non gli interessa; vorrebbe la bigliettazione integrata, vorrebbe la promozione integrata e orari compatibili. Lavorare sul sistema museale, anche e non solo su quello statale: questo è il compito dei poli museali.

perché il Louvre è dodici volte più grande degli Uffizi che sono al massimo della capienza e sono a numero chiuso, quindi non possono crescere come numero di presenze. Se guardiamo, invece, il dato complessivo, l'Italia è assolutamente il primo Paese in quanto a numero di visitatori,

verrà restituito alla città, con una cerimonia di inaugurazione, il restauro dell'esterno, grazie ai finanziamenti dell'impresa. I lavori proseguiranno con l'intervento sugli ipogei, a cui si aggiungono le risorse pubbliche - pari a 18 milioni di euro per il restauro e la ricostruzione dell'arena, che secondo me costituisce un grande passaggio di valorizzazione del Colosseo. Quanto al centro servizi, in

sono state stanziate per i piccoli interventi di manutenzione, ma per questo settore ci sono altre risorse, che sono state reintrodotte nella legge di stabilità dell'anno scorso. Il mio Ministero, quando sono arrivato, aveva 35 milioni

Penso che i cammini siano un veicolo formidabile per il turismo sostenibile e la valorizzazione delle parti meno conosciute del nostro Paese. E penso che abbiamo fatto una scelta conseguente a questa dichiarazione di principio,

delle strutture recettive, al fine di colmare quel ritardo strutturale che c'è, sia nel pubblico che nel privato, in materia di offerta digitale del turismo, che è il settore che più di tutti è entrato nel mondo digitale.

abbiamo cambiato la ragione sociale, è diventato un ente pubblico economico, ne abbiamo modificato la *governance*, tutto il personale ha scelto di restare nel settore pubblico, quindi la nuova *governance* dell'ENIT sta assumendo attraverso delle procedure di selezione delle persone che siano in grado di stare nel mondo competitivo del turismo. Naturalmente i cambiamenti non si fanno

sono soddisfatto e sono contento che il Ministro si sia convertito sulla via del Colosseo. Visto che noi abbiamo firmato la convenzione con Gianni Letta e Silvio Berlusconi, spero che il ministro Franceschini li menzioni domani quando verranno restituiti i restauri dei prospetti meridionali e settentrionali del Colosseo e degli ambulacri. È un restauro integrale, imponente, importante; tutti gli atti sono firmati da Silvio Berlusconi; fu fatta una convenzione con la Tod's SpA di Diego Della Valle. Ricordiamolo ogni tanto.

che lo avevo fatto perché non avevo trovato il palazzinaro di Roma, perché immaginavo che i grandi costruttori, che sono il pilastro dell'economia romana, si rendessero disponibili per restaurare un monumento: non era una scarpa, ma un monumento. Mi hanno accusato di voler cartonare il Colosseo. È stato cartonato? No, perché Diego Della Valle andava in Cina, in Brasile ed era lo *sponsor* unico del Colosseo. Questo era

che il Governo sta dedicando al settore dei beni culturali e monumentali in Italia. Io continuo ad avere un tarlo in testa, che è quello di percorrere la strada della

trinomio tra cultura, turismo e innovazione come fattore strategico per promuovere lo sviluppo del Paese, anche nell'ottica di ridurre il

io mi dichiaro soddisfatto della risposta del Ministro. Ritengo che il ministro Franceschini abbia fatto in passato un ottimo lavoro e sono convinto che anche in futuro farà delle cose molto importanti e innovative per la cultura e il turismo in Italia.

e francigeno, che non hanno niente da invidiare a Santiago di Compostela. La via Francigena passa anche nella mia Aulla, dove c'è il Santo protettore. Qui hanno scoperto le spoglie mortali del Santo della via Francigena, un evangelizzatore nato nel Medio Oriente che ha fondato un importante ordine cistercense in Francia. Ieri ero con il suo sottosegretario Dorina Bianchi a Viterbo.

Sono soddisfatto per quanto riguarda la cifra stanziata dal CIPE. Per questo ha assolutamente ragione. Non sono soddisfatto per le non politiche turistiche che stiamo facendo in questo momento in Italia. Non lo dico io, ma i colleghi dei vari *tour operator*, delle agenzie di viaggio e tutti coloro che operano nel settore. A me duole leggervi quattro righe: «L'Italia, pur avendo un patrimonio turistico unico al mondo (arte, storia, cibo, mare, montagna e città, solo per citare alcune delle attrattive), sta purtroppo perdendo terreno: l'offerta non si è evoluta, la promozione all'estero è poca cosa, le istituzioni non hanno una politica di promozione ben delineata e la presenza sul *web* è molto deficitaria. Il Belpaese è ormai scivolato al sesto posto» - avevo ragione

Adoro il vostro ottimismo renziano; il problema è che il nostro settore del turismo - lo ripeto ancora una volta - sta aspettando delle risposte e, in questo caso, non c'è competenza per quanto riguarda il mondo del turismo. Signor Ministro, l'ho ascoltata con attenzione e interesse. Lei ha effettivamente, come sempre ha dimostrato, una visione ampia e complessiva del settore. Questo la grava di ulteriori responsabilità, nel senso che, all'interno del Governo, deve far intendere che questo è un settore su cui assolutamente occorre investire ancora di più. Il turismo e, particolarmente, quello culturale può essere per lo sviluppo e può produrre nuovi posti di lavoro, specialmente per quella disoccupazione intellettuale che tanto ci preoccupa. In merito alla detassazione di cui ho chiesto nel mio intervento, ritengo che il Governo debba fare ancora di più se vuole cogliere i frutti di uno sviluppo complessivo.